Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, rappresentante del Governo, iniziamo oggi questo importante Atto Senato 411, che va a porre mano al decreto legislativo

urge la necessità di adeguare il codice della proprietà industriale, inteso anche come proprietà intellettuale (per quanto concerne i brevetti),

con questa modifica, che poi diventa un'implementazione legislativa, si adegua e si vanno a porre modifiche importanti, principalmente attraverso l'articolo 1 e l'articolo 3. L'articolo

da rischi di usurpazione e imitazione, che sappiamo essere frequenti nel mercato internazionale. Per citarne alcuni, ricordiamo il "parmesan" piuttosto che il "prosek". Sono tentativi malvestiti di appropriarsi di marchi importanti, frutto di generazioni di lavoro, ma soprattutto di grandissima professionalità, che indubbiamente fanno la differenza e che dobbiamo assolutamente

su quello che è, invece, il rapporto che si instaura tra l'inventore e l'ente con cui lo stesso lavora, spesso istituti di ricerca, università o anche datori di lavoro.

che hanno implementato, da un punto di vista legislativo, il precedente decreto. Ebbene, è stato un lavoro importante, già iniziato nella precedente legislatura, che si pone come obiettivo quello di essere

quindi tutti per il proficuo lavoro svolto e mi accingo ora a leggere la relazione già allegata agli atti, per toccare in maniera specifica i vari punti. Il disegno di legge Atto Senato 411 si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La componente 2 della Missione 1 è volta a perseguire la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo. In questa area di intervento si inserisce la misura relativa alla riforma del sistema della proprietà industriale del PNRR, con scadenza entro il terzo trimestre del 2023. Gli obiettivi della riforma sono: rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale; incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle piccole e medie imprese; facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo, nel contempo, un equo rendimento degli investimenti.

La sua implementazione legislativa prevede la modifica del già citato decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005, cioè il codice della proprietà industriale, per disciplinare almeno la revisione del quadro normativo, per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure, il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenza, l'agevolazione del trasferimento di conoscenze, il rafforzamento della promozione dei servizi innovativi. Il disegno di legge reca quindi specifiche norme finalizzate alla realizzazione dei predetti obiettivi. Un identico testo era già stato già stato presentato in Senato nella XVIII legislatura, come prima accennavo, quale collegato alla manovra di finanza pubblica, a seguito di una consultazione pubblica svolta dall'allora Ministero dello sviluppo economico, e ne era stato avviato l'esame in 10a Commissione, non concluso per la fine anticipata della legislatura. Nell'attuale legislatura, la 9a Commissione ha svolto una approfondita discussione dopo un nutrito ciclo di audizioni con gli operatori del settore. Venendo all'articolato, per rafforzare la tutela connessa ai diritti della proprietà industriale e al sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, il disegno di legge prevede, in di rafforzare la tutela delle denominazioni di origine protetta e le indicazioni protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose e in particolare di quelle prive di un consorzio di tutela riconosciuto, riconoscendo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la legittimazione a proporre opposizione dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, alla registrazione di marchi identici o simili a tali denominazioni e indicazioni di origine privi di consorzio di tutela, ai sensi di ribaltare l'approccio del cosiddetto *professor's privilege*, previsto nell'attuale CPI - quindi, come detto, il rapporto cambia - portando la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca nelle strutture universitarie alla struttura di appartenenza e, solo nel caso in cui quest'ultima non intenda avvalersene, al ricercatore. avvalersene, al ricercatore. A tale ultimo riferimento, in 9a Commissione sono stati apportati importanti modifiche al testo originario del Governo, frutto dei numerosi rilievi avanzati durante le audizioni. In sintesi, sono stati chiariti i rapporti tra l'inventore e la struttura di appartenenza in tutte le fasi del procedimento e precisate le tempistiche per la domanda di brevetto. Un'ulteriore modifica ha riguardato la disciplina dei diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca: nel testo originario era fissata una percentuale di remunerazione per l'inventore non inferiore al 50 per cento degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico dell'invenzione. Facevo non a caso riferimento prima agli articoli 64 e 65 del precedente decreto legislativo. Quindi abbiamo effettivamente lasciato libertà di rapporto tra l'inventore e l'istituto con cui lo stesso ha rapporti di lavoro. La Commissione ha scelto infatti di demandare la fissazione di tale soglia agli accordi contrattuali tra le parti, redatti sulla base di linee guida adottate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca. di chiarire i rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano, stabilendo che, qualora per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore siano stati concessi un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi medesimi data di deposito e di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo, come stabilito dall'articolo 5. Si prevede, inoltre, di garantire la protezione temporanea a disegni e modelli esposti in fiere, dell'articolo 2, la possibilità di ottenere il sequestro di prodotti contraffatti esposti nelle stesse, ai sensi dell'articolo 22, nonché di ampliare le ipotesi in cui è possibile agire in via amministrativa per chiedere la nullità di marchi,

che devono essere resi pubblici mediante trascrizione ai fini dell'opponibilità verso i terzi (articolo 26); rafforzare il controllo preventivo sulle domande di brevetto utili

8); consentire di agire in sede amministrativa per l'annullamento della registrazione di marchi lesivi dell'immagine della reputazione dell'Italia (articolo 26). Con riferimento alla semplificazione delle procedure, si richiama: l'introduzione del cosiddetto principio *first to file*, che consente la conservazione della data di deposito della domanda di brevetto anche quando il pagamento dei diritti di deposito sia stato effettuato in data successiva al deposito stesso (articolo 7); la possibilità di accedere al sistema di deposito telematico dell'UIBM previo accertamento dell'identità digitale al riguardo, la 9a Commissione ha introdotto precisazioni ulteriori circa i tempi per effettuare la richiesta di trasmissione degli atti dei documenti originali. prevista la possibilità di utilizzare, dinanzi al medesimo ufficio in sede di rivendicazione delle priorità, in alternativa alla copia della domanda, codici identificativi della stessa presso banche dati detenute da altri soggetti (articolo 13); 13); la razionalizzazione e l'armonizzazione degli importi dell'imposta di bollo, che amplierebbe, secondo le valutazioni del Governo, le possibilità di utilizzo del bollo digitale (articolo 31). Una serie di norme è poi rivolta allo snellimento della fase procedimentale, di esame della richiesta di registrazione, modifica o trasferimento di un titolo. Tra esse si segnalano: la soppressione della Commissione consultiva attualmente prevista nella procedura di registrazione di privativa di nuova varietà vegetale con il riconoscimento al solo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del potere di esprimere parere vincolante sulla registrazione (articolo 14); la riduzione, da quaranta a trenta, del numero dei giorni minimi intercorrenti tra l'udienza di trattazione presso la Commissione ricorsi e la relativa convocazione delle parti (articolo 10); l'opponibilità ai terzi degli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero che modificano i diritti inerenti a una domanda o a a un brevetto europeo, direttamente per effetto dell'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti (articolo 11); da due a quattro anni della durata in carica della Commissione ricorsi, in modo da limitare, secondo l'intenzione del Governo, gli oneri amministrativi derivanti dalla procedura di rinnovo (questo è indubbiamente un buon passaggio per ridurre i tempi); In proposito, il testo originale del Governo prevedeva la presenza solo di due consulenti in proprietà industriale abilitati, mentre la 9a Commissione ha scelto di riportare tale numero a come attualmente previsto. È poi prevista una nuova articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione (articolo 25). Quanto alla revisione del quadro normativo in materia di proprietà industriale, al fine di renderlo più chiaro, e dunque meglio applicabile, si evidenziano: l'aumento della sanzione amministrativa - attualmente irrisoria per chi appone su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto,

l'intervento sulla proroga dei termini dei procedimenti presso l'UIBM, la cui durata massima viene ora più chiaramente indicata in sei mesi dalla scadenza del termine per cui viene chiesta chiesta (articolo 16); l'allungamento a un anno dei termini delle istanze di reintegrazione la precisazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e del brevetto per modello di utilità (articolo 20); gli interventi finalizzati ad abrogare esplicitamente le previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione (articolo 21). Relativamente allo sviluppo delle abilità e competenze e al trasferimento delle conoscenze, viene introdotta nel codice la disciplina degli uffici di trasferimento tecnologico (UTT), presso le università, gli enti pubblici di ricerca e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), funzione di raccordo con le imprese (articolo 4). Tale previsione è anche funzionale al rafforzamento delle imprese e degli enti di ricerca. In ordine alla promozione di servizi innovativi, ivi inclusa la loro digitalizzazione, il disegno di legge prevede la soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea da parte di uffici o enti all'UIBM e la semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico, sempre presso l'UIBM l'UIBM (articolo 12). La possibilità di utilizzare - in sede di rivendicazione della priorità di un deposito di una domanda per ottenere un titolo di proprietà industriale codici identificativi presenti in banche dati presso cui l'ufficio può direttamente verificare il contenuto di documenti senza che questi debbano essere depositati (articolo 13). Infine, in 9a Commissione si è intervenuti per sopprimere l'articolo 29 del testo originario, non essendo necessari interventi attuativi per adeguare il codice alle novelle apportate dal disegno di legge in esame.

Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, le modifiche sottoposte oggi alla nostra attenzione sono un ulteriore passo nel processo di attuazione degli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ancora una volta i fatti dimostrano che l'attuale Governo rispetta gli impegni assunti con i cittadini, garantendo lo sviluppo e la crescita del Paese. Ci tengo fin da subito a ringraziare il ministro Urso per il lavoro svolto che, riprendendo il percorso avviato dal precedente Governo, è stato arricchito attraverso il confronto con la Commissione parlamentare competente - quella della quale sono membro - consentendoci oggi, dopo un lungo, ma serrato esame, di discutere e votare un testo migliorato, riscontrando appieno gli obiettivi di rafforzamento della competitività del sistema Paese

perché dovremmo essere sempre orgogliosi di quello che siamo stati nella storia del mondo. Sono modelli per noi e per le future generazioni. In questo quadro la tutela delle idee, dei marchi e dei prodotti dell'ingegno è fondamentale perché agisce da stimolo per l'innovazione, spingendo la ricerca e consentendo salvaguardia della qualità. Basti pensare che le industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale generano nel nostro Paese oltre il 52 per cento del PIL e contribuiscono al 28 per cento dell'occupazione, dati questi molto più alti della media europea. Tra le misure che ci stanno particolarmente a cuore e che hanno trovato accoglimento in questo disegno di legge c'è, in primo luogo, il rafforzamento della tutela delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni agricole alimentari e vinicole, che vede anche l'attribuzione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare delle foreste del potere di proporre opposizione alla registrazione di marchi identici o simili a tali denominazioni. Con questa misura rafforziamo il nome dell'Italia, dei suoi luoghi e dei suoi prodotti caratteristici, che ovunque nel mondo sono sinonimo di qualità e per questo troppo spesso vittime di usurpazione. Siamo d'accordo con il ministro Lollobrigida, che in queste ore ha detto una cosa sacrosanta, cioè che qualità nel mondo è sinonimo di Italia. Positivo è anche il superamento del *professor's privilege*, che permetterà di fatto una reale valorizzazione del lavoro d'*équipe* e del fondamentale contributo che i ricercatori inseriti in contesti universitari ricevono dalla struttura di appartenenza. Sul punto, peraltro, la Commissione ha raggiunto un ottimo equilibrio rispetto alla proposta iniziale, promuovendo il principio dell'autonomia negoziale delle parti piuttosto che quello dell'imposizione normativa. Particolarmente importanti sono poi quegli interventi volti alla semplificazione delle procedure e alla loro digitalizzazione, che consentono un confronto più facile degli interessati con la pubblica amministrazione. l'introduzione del codice della disciplina degli uffici di trasferimento tecnologico, istituiti presso le università e gli enti pubblici di ricerca, è particolarmente rilevante. Tali uffici promuoveranno infatti un raccordo con le imprese, garantendo lo sviluppo delle abilità e delle competenze, oltre al trasferimento in concreto delle nuove conoscenze. Da ultimo, voglio citare anche l'articolo 26, che vieta esplicitamente la registrazione di marchi lesivi dell'immagine dell'Italia, come ho poc'anzi detto, e che dimostra l'attenzione del Governo e di questa maggioranza alla protezione della reputazione del nostro Paese e talvolta dovremmo anche occuparci del vilipendio, che spesso e volentieri, soprattutto nella mia terra, viene fatto del nostro Paese e dei simboli che lo rappresentano. Concludo, Presidente, ricordando come questo provvedimento porti a compimento un lungo percorso già avviato nelle precedenti legislature e che ha ricevuto l'apprezzamento da parte delle categorie produttive mettendosi in tal modo in linea di continuità con il processo di ammodernamento del Paese che stiamo portando pervicacemente avanti. Il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia -Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE per questi motivi voterà convintamente a favore di questa proposta, che ci permette anche di rispettare i tempi che ci siamo dati per l'attuazione delle misure del PNRR, come ha sostenuto il ministro Fitto, di cui questo provvedimento è e resta una pietra miliare.

la riforma del sistema di proprietà industriale è prevista dalla missione 1 del PNRR. Si tratta di un tema fondante la nostra economia e particolarmente importante perché tocca le eccellenze delle nostre imprese non solo del settore manifatturiero ma anche di quello agroalimentare. potenziarlo e rafforzarlo significa aumentare la competitività del sistema Paese, incentivare l'uso della proprietà industriale da parte di piccole e medie imprese, tutelando la nostra straordinaria creatività. Il Governo Draghi fu il primo ad approvarlo nell'aprile dello scorso anno in una formulazione identica a quella ripresentata in quest'Aula dal nuovo Esecutivo. Le modifiche introdotte in Commissione non ne hanno stravolto la *ratio*, quindi non abbiamo difficoltà a confermare la nostra condivisione relativamente alle misure contenute nel disegno di legge e non facciamo fatica ad auspicare che ci possa essere un rapido passaggio parlamentare.

nel PNRR, di un'occasione straordinaria. Abbiamo quindi, come sempre, un atteggiamento di opposizione responsabile. Il giudizio positivo

In Commissione si è svolto un dibattito che ha messo in rilievo la necessità e l'opportunità di approvare questo provvedimento. Peraltro, è stata sottolineata una volta di più la centralità e il protagonismo della ricerca come elemento essenziale della nostra economia. Le imprese italiane, diversamente dal passato, fanno un utilizzo accorto e investimenti importanti nell'ambito della ricerca, che infatti sono quasi raddoppiati negli ultimi vent'anni anche grazie alle misure di Industria 4.0. Dall'ingegneria elettrica alle tecnologie medicali, dalle biotecnologie alla meccanica, cresce l'investimento in ricerca e la consapevolezza delle imprese di quanto

costituiscono un *asset* fondamentale della nostra economia e le misure contenute in questo disegno di legge vanno nella giusta direzione. Ovviamente molto resta ancora da fare. C'è un tema molto importante che riguarda la tutela delle nostre eccellenze e la lotta all'*italian sounding*; penso in particolar modo all'industria agroalimentare. C'è ancora moltissimo da fare per tutelare gli investimenti in qualità delle nostre imprese, però questo provvedimento va nella giusta direzione. Sottolineo l'articolo 65 del codice della proprietà industriale, perché con la norma in questione i diritti nascenti da un'invenzione non spetteranno più esclusivamente all'inventore, ma alla struttura di appartenenza; è stato un elemento di dibattito, quello del superamento del *professor's privilege*, però è un fatto importante che ci allinea alla normativa europea. Sempre nell'ottica di rafforzare i ponti fra ricerca pubblica e imprese, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici e gli IRCCS potranno dotarsi di un ufficio di trasferimento tecnologico: questo è un fatto molto importante, perché quell'ufficio avrà la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale anche attraverso la promozione di una collaborazione fra le imprese. Insomma, il disegno di legge in questione rafforza anche la tutela delle indicazioni geografiche e le denominazioni di origine italiana e unionista, in favore della competitività dell'industria del *food*, di primario interesse interesse per il *made in Italy*. Lo fa estendendo il divieto di registrazione come marchi di impresa a tutti i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protetta in base alla normativa statale e unionale, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte. E lo fa anche includendo esplicitamente, tra i soggetti legittimati a proporre opposizione a una domanda o registrazione di marchio, di marchio, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quale autorità nazionale competente per le DOP, le IGP e le IG agricole, alimentari e dei vini, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto. Trovo che anche questa sia una via istituzionale corretta per difendere la qualità delle nostre produzioni. Il provvedimento contiene anche misure, non meno importanti ma più tecniche, di semplificazione e di digitalizzazione di alcune attività svolte presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Viene estesa la durata in carica della commissione dei ricorsi da due a quattro anni, vengono ridotti i termini per la discussione dei ricorsi, viene eliminato l'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea, viene semplificata la modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico. Naturalmente la tutela del *made in Italy* non può fermarsi qui; occorrono anche interventi strutturali per permettere al nostro apparato industriale di tenere il passo con le transizioni in corso e di esserne protagonista. Accanto alla sottolineatura, che facciamo ancora una volta, per il ripristino di Industria 4.0, annuncio il voto favorevole di Azione-Italia Viva a questo provvedimento.

al nostro esame - come è già stato detto - era stato presentato dal Governo Draghi. Il Governo Meloni lo presenta in un testo identico. Nella scorsa legislatura non fu possibile approvarlo, anche perché è finita prematuramente, come tutti sappiamo. Esso fa parte delle riforme legate al PNRR e quindi è fondamentale la sua approvazione. Va ricordato che il Governo Meloni e il Ministero delle imprese e del *made in* *Italy*, prima di presentare il disegno di legge, hanno elaborato le linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale 2021-2022; e bene hanno fatto a sottoporle a consultazione pubblica prima di adottarle. L'esito della consultazione ha evidenziato che l'attuale sistema rende difficoltoso accedere agli strumenti di difesa della proprietà industriale ed è connotato da procedure articolate e complesse, rispetto alle quali sono stati richiesti appositi interventi di semplificazione e digitalizzazione. Gli obiettivi di questa riforma del codice della proprietà industriale saranno: rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale, incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale (in particolare da parte delle piccole e medie imprese), facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti, garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale e rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale (cosa della quale abbiamo davvero bisogno). La riforma deve entrare in vigore entro il terzo trimestre 2023, sempre secondo gli accordi sul PNRR. L'obiettivo pratico della stessa è quello di finanziare almeno 254 progetti aggiuntivi, sostenuti da opportunità di finanziamento connesse alla proprietà industriale e destinate a imprese e organismi di ricerca entro il quarto trimestre dell'anno 2025. La ricaduta pratica sul mondo delle imprese ha diverse implicazioni: la revisione del quadro normativo per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure, il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze, l'agevolazione del trasferimento di conoscenze, il rafforzamento della promozione dei servizi innovativi. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2021 sono state ben 186.000 le domande di titoli di proprietà industriale e di istanze ad esso collegate presentate in Italia. Si tratta di circa 50.000 brevetti, di cui 9.000 italiani, mentre 36.000 sono convalide di brevetti europei che che devono essere registrate in Italia. Ecco perché la necessità di inserire il provvedimento nell'ambito delle riforme chieste dall'Europa. Quasi 71.000 sono state le domande di deposito di marchio, di cui 48.000 di primo deposito, e 1.800 le domande di opposizione di marchio a tutela del proprio. E sono ben 218 i marchi storici di interesse nazionale che hanno più di cinquanta anni tutelati nel solo 2021; quasi 25.000 i disegni e i modelli contenuti nelle oltre mille domande nel 2021. Un quadro, quindi, colleghi, a tutela delle nostre imprese e delle *start up* innovative, che hanno appunto un marchio ed un brevetto dal quale muovere la propria attività, spesso molto innovativa. poi ricordato che il quadro normativo nazionale si inserisce in un quadro europeo e internazionale di protezione dei diritti della proprietà intellettuale. Il disegno di legge, quindi, nei suoi 32 articoli va a modificare ed integrare gli articoli del codice della proprietà industriale. Innanzitutto, si introduce il divieto di registrazione come marchi di segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine protetta, in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia e l'Unione europea sono parte. E sappiamo che l'Italia ha una grande necessità di tutelare le sue più di 1.500 DOP, IGP e IG, cioè quei prodotti tipici italiani che spesso vengono copiati con nomi simili, ma con contenuti assai differenti rispetto all'originale. Viene inoltre inserito nel codice un nuovo articolo, che prevede la protezione temporanea dei disegni e dei modelli, che figurano in una esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o di uno Stato estero con il quale si abbiano accordi di reciprocità di trattamento. Come già è stato detto, l'approccio in vigore sulla titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle università o degli enti pubblici di ricerca. Ora si prevede che i diritti nascenti dall'invenzione spettino alla struttura di appartenenza dell'inventore, a meno che la stessa struttura chiaramente non ne abbia interesse. Sempre nell'ambito universitario, viene prevista la possibilità di dotarsi di un ufficio di trasferimento tecnologico, al fine di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni tra le università e le imprese. Non devo sottolineare come sia importante che si crei un legame più forte, così forte, tra l'universo della ricerca e il mondo delle imprese. Viene poi prevista la coesistenza tra brevetto europeo e brevetto italiano. Si prevede il rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato. Sono rimodulati sistema e tempi dei ricorsi sulla titolarità dei diritti, così come cambia il livello delle sanzioni. A tutela del nostro Paese, viene introdotto un nuovo motivo per il quale può essere chiesta la nullità del marchio, consistente nella registrazione di parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia. Insomma, una serie di modifiche puntuali e tecniche al codice della proprietà industriale, che vanno incontro alle esigenze rappresentate dagli *stakeholder,* rappresentate anche durante l'esame puntuale della 9ªCommissione, che ha lavorato al testo in sede redigente. Un provvedimento, quindi, colleghi, che ci si augura possa contribuire non solo ad aumentare il numero dei brevetti registrati, ma anche ad avere maggiori certezze nella risoluzione delle controversie e ad utilizzare al meglio i canali digitali, a tutela delle nuove idee delle imprese italiane e del *made in Italy*. Per queste ragioni, Forza Italia vede con favore l'approvazione di questo provvedimento e quindi voterà favorevolmente.

da più parti, questo disegno di legge, con cui si modifica l'attuale codice di proprietà industriale, si incasella nel più generale obiettivo previsto dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La componente 2 di detta missione, infatti, è volta a perseguire la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo. Proprio in quest'area di intervento si inserisce la misura relativa alla riforma del sistema della proprietà industriale, vista come un aspetto cruciale per la tutela delle idee, dello sviluppo lavorativo e di quanto venga generato dall'innovazione e per assicurare un vantaggio competitivo a chi si sia attivato in questo ambito. Un testo questo che è stato presentato nelle ultime battute della precedente legislatura e che non è giunto al termine della trattazione a seguito della caduta del Governo e delle elezioni anticipate. Ora il medesimo schema, come sappiamo bene, proprio per rispettare le tempistiche del PNRR, deve essere approvato, insieme agli atti attuativi, entro il terzo trimestre del 2023. Un obiettivo temporale, quest'ultimo, che si aggiunge alle finalità che l'azione normativa vuole perseguire, vale a dire la revisione della vigente disciplina per la semplificazione delle procedure, il rafforzamento della tutela dei diritti di proprietà industriale, il perfezionamento dello sviluppo di abilità e competenze, l'agevolazione del trasferimento di conoscenze, la promozione dei servizi innovativi e il consolidamento del ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale. Il nostro contributo rispetto a questo impulso normativo, di iniziativa governativa, è stato del tutto costruttivo, a partire dal numero di emendamenti proposti, che è stato ridotto e orientato esclusivamente ad un miglioramento dei contenuti, anche sulla base di quanto è emerso durante il ciclo di audizioni in Commissione. L'azione che abbiamo messo in campo, quindi, è stata soprattutto mirata a proteggere il patrimonio agroalimentare italiano, quale volano dell'economia ed esempio emblematico della libera concorrenza e del mercato. Abbiamo poi cercato di tutelare maggiormente il consumatore, affinché proceda ad acquisti salutari e sicuri, specialmente per quanto riguarda la corretta individuazione della provenienza e l'esattezza delle informazioni abbiamo inteso difendere i nostri segni distintivi per il comparto agricolo e rurale, che è contemporaneamente custode di storia, cultura e tradizione. tal proposito, prendendo spunto dal rilievo del Comando dei carabinieri per la tutela agroalimentare, abbiamo proposto un innalzamento degli importi della sanzione amministrativa relativa al caso in cui si appongano indicazioni su un prodotto che tendono a far credere che lo stesso sia protetto da un brevetto, oppure a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato. Questo intervento ha una chiara efficacia deterrente, proprio per scoraggiare quei comportamenti che, fino ad ora, non fanno altro che generare confusione nei consumatori, alimentando per assurdo un generalizzato clima di sfiducia anche nei confronti di quegli imprenditori onesti che invece agiscono nel pieno rispetto delle regole. L'apporto emendativo è stato parzialmente accolto: dico «parzialmente» perché la forbice degli importi sanzionatori da noi proposta era superiore rispetto a quella poi effettivamente approvata. Con un Governo che vanta tra i propri Dicasteri quello per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste ci saremmo aspettati che l'emendamento che abbiamo presentato sul rafforzamento del contrasto all'*italian sounding* fosse approvato, ma così purtroppo non è stato. In sostanza avevamo proposto di definire in maniera chiara e inequivocabile le regole a cui si devono attenere gli operatori che compiono una serie di attività nella catena commerciale riguardanti i prodotti agricoli o alimentari che provengono da un Paese diverso da quello di vendita. Questi soggetti devono indicare in maniera precisa, a caratteri ben chiari, il Paese o il luogo di fabbricazione o di produzione del prodotto che viene messo in vendita. Questo perché le indicazioni sono l'unica bussola a disposizione del consumatore nel *mare magnum* degli acquisti ed è importante che non si creino dubbi o errori sull'effettiva origine dei prodotti stessi. Sempre in tema di *italian sounding* e di salvaguardia delle eccellenze che contraddistinguono l'Italia a livello internazionale, abbiamo proposto che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* notifichi ai consorzi di tutela interessati e alla parte lesa i casi di pirateria relativi alla contraffazione o all'alterazione dei marchi agroalimentari. Quanto detto, infatti, serve ad evitare che tutti i soggetti parzialmente coinvolti continuino a correre il rischio di essere all'oscuro di quanto sta accadendo ai loro danni o che magari giungano a conoscenza della lesione subita quando ormai gran parte delle azioni risolutive sono state oltrepassate dal fattore tempo. L'*Italian sounding*, infatti, riguarda quasi sempre alimenti etichettati ingannevolmente, con diciture, simboli o immagini che richiamano valori legati al contesto paesaggistico e culturale italiano, ingenerando in chi compra l'equivoco che l'intera filiera si sviluppi nel nostro Paese e che le materie prime agricole utilizzate nel processo di trasformazione abbiano origine in Italia. Questa pratica ingannevole è diffusissima all'estero, in quanto non sempre il consumatore straniero riesce a distinguere un vero prodotto italiano da uno che suona italiano. Tale fenomeno, tuttavia, si sta espandendo anche a livello interno, con preoccupanti riverberi per la filiera del *made in Italy*, perché sta assumendo delle dimensioni spropositate. Solo nel 2022, grazie all'intervento investigativo dell'Arma dei carabinieri, sono state scoperte ben 3,4 milioni di euro di frodi agroalimentari e sequestrate 5.400 tonnellate di prodotti non sicuri. Ciò per dire che, se riusciamo a introdurre dei correttivi in tutte le fasi che si collegano alla problematica, anche per gli aspetti di interesse contenuti nel codice della proprietà industriale, possiamo certamente contribuire ad alleviare una piaga che affligge non solo il settore primario, ma anche quello dell'industria agroalimentare, dell'*export* e dell'intero tessuto produttivo interno. Con riguardo all'istruttoria eseguita dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la registrazione di un marchio che afferisce a produzioni agricole con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, con le corrispondenti abbreviazioni DOP o IGP, sarebbe stata auspicabile l'acquisizione preliminare di un parere da parte dei Consorzi di tutela coinvolti, ove presenti: un rilievo, questo, emerso sempre grazie al contributo del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare e che abbiamo prontamente recepito attraverso la stesura di una proposta emendativa. La finalità, come al solito, è stata assolutamente di buon senso: evitare futuri contenziosi e limitare preventivamente richieste indebite di registrazione di marchi che lederebbero la proprietà industriale. In generale, linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale rappresentano un pacchetto di notevole importanza e valenza strategica per la protezione e l'incentivazione dell'innovazione, che costituisce sempre di più un fattore cruciale di sviluppo per la nostra società. La norma chiarisce anche i diritti nascenti dall'invenzione, che saranno disciplinati da accordi contrattuali tra le parti, tenendo conto di linee guida che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* dovrà emanare sessanta giorni dall'approvazione del disegno di legge. Inoltre, si mette un punto fermo sulla possibile coesistenza del brevetto italiano, per una stessa invenzione e medesimo inventore, con un eventuale brevetto europeo. Sulla base di queste premesse, è nostro dovere non rallentare l'*iter* del PNRR, già gravato da una gestione di questo Governo che non si può definire certamente attenta alle scadenze. La nostra è un'opposizione acritica e ragionevole, ma costruttiva, perché orientata al solo ed esclusivo interesse della collettività. Per questa ragione annuncio, a nome del mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle, il voto favorevole a questo disegno di legge.

Non solo il cibo italiano, la dieta mediterranea ed il vino, di cui siamo i primi produttori al mondo, con buona pace delle illusioni dei cugini di Francia; *made in Italy* è sinonimo di eccellenza nella moda, nell'industria, nell'artigianato, nell'automobile. Ogni settore esprime l'estro del genio e il senso del bello italiano. Il disegno di legge che ci apprestiamo a votare oggi si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dalla missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e si pone, in coerenza con il Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'Unione europea, adottato dalla Commissione europea lo scorso 25 novembre, a tutelare e nobilitare il *brand* del *made in Italy*.

rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale, incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare, da parte delle piccole e medie imprese, il vero tessuto economico del nostro Paese; facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione; garantire nel contempo un equo rendimento degli investimenti; garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale. La tutela del patrimonio Italia resta la priorità di questo Governo, ed è per questo che il disegno di legge in oggetto rappresenta una riforma attesa dall'industria, utile a modernizzare aspetti essenziali del diritto della proprietà industriale. È necessario, allora, Presidente, ricordare e sottolineare che in Italia le industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale generano oltre il 52 per cento del Prodotto interno lordo e contribuiscono al 28 per cento dell'occupazione. Parliamo di *performance* nettamente superiori alla media europea. Troppo spesso dimentichiamo che, dietro i beni immateriali, come i brevetti, il *franchising*, l'avviamento, marchi, nomi commerciali, persino *software*, si celano il lavoro, l'impegno e l'inventiva di tante persone, di tanti italiani, i quali costituiscono il reale valore economico e produttivo di ogni impresa il principale fattore di competitività di un Paese a livello globale. Questo per l'Italia ha un valore nettamente superiore rispetto a tutti gli altri Paesi del mondo: nessuno ha il nostro afflato e la nostra inimitabile inventiva. infatti il contributo delle imprese italiane a questo campo è centrale, sia guardando agli investimenti in innovazione sia guardando agli investimenti soprattutto in attività e inventiva. Negli ultimi vent'anni l'investimento in ricerca e sviluppo delle imprese italiane è quasi raddoppiato, con un'accelerazione nell'ultimo triennio, nonostante la crisi economica, di quasi il quattro per cento nel 2022 rispetto all'anno precedente. Gli investimenti pubblici in innovazione, purtroppo, sono rimasti sostanzialmente stabili, contro una media europea che è quasi il doppio della nostra, e questo non è un dato da tenere in secondo piano. Per quel che concerne poi l'aspetto brevettuale, le imprese italiane sono all'avanguardia: nel 2021 abbiamo registrato un incremento delle domande di brevetto europeo depositate del 6,5 per cento rispetto all'anno precedente, e ancora una volta si è trattato di un risultato superiore alla media degli altri Paesi: più 2,8 per cento. Esprimiamo soddisfazione per l'approvazione di una nostra proposta di modifica dell'articolo 65 del codice in materia di titolarità delle invenzioni. In particolare, quando un'invenzione industriale viene fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro con una università, anche non statale ma legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca, un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto l'autore. L'obiettivo che si intende perseguire è quello di favorire i processi di trasferimento tecnologico dal mondo delle università a quello delle imprese, ribaltando l'approccio fino ad oggi in vigore relativamente alla titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca. È stato poi approvato all'unanimità l'ordine del giorno, sottoscritto da molti senatori del Gruppo Lega, per il riconoscimento della centralità del nostro Paese nel panorama brevettuale europeo, con la richiesta di assegnazione alla città di Milano della sede della terza divisione centrale del tribunale unificato europeo dei brevetti. Ringrazio la Commissione perché è un risultato molto importante e di sostegno a questo. Grazie al provvedimento in discussione, finalmente inizierà un giro di vite sui marchi evocativi e usurpativi dei prodotti DOP e IGP. È una delle novità presenti nel disegno di legge che modifica il codice della proprietà industriale. Contrastare ogni utilizzo improprio di un patrimonio che rappresenta un vanto e dà un importante contributo all'economia nazionale significa infatti tifare per la crescita globale del nostro Paese. La modifica al codice della proprietà industriale nel primo articolo riprova e chiarisce che la protezione è da intendersi in senso estensivo, vietando la registrazione di marchi, e anche di servizi evocativi o usurpativi, di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta, e rafforza il controllo preventivo rispetto al deposito relativo alle domande di brevetto potenzialmente utili per la difesa del Paese. Quello che stiamo facendo è difendere quell'eccellenza italiana da sempre riconosciuta nel mondo come fondata sui principi del bello, del benfatto e della qualità assoluta. Da tempo assistiamo ad una delegittimazione dei prodotti italiani portata avanti mediante vari tentativi mal riusciti supportati dall'Unione europea. Purtroppo a lungo l'abbiamo subita passivamente: dal "prosek" al "parmesan" sono innumerevoli i casi di imitazione delle eccellenze italiane nel mondo che, sfruttando il fenomeno dell'*italian sounding,* inducono i consumatori a considerare italiani prodotti in realtà realizzati all'estero, di pessima qualità, che nulla hanno a che fare con le eccellenze del nostro Paese, sottraendo alla nostra economia, come ben sappiamo, circa 130 miliardi di esportazione ogni anno. Pensiamo poi a regole imposte dall'Unione europea, come ad esempio quella sull'etichettatura fuorviante dei vini o il nutri-score*,* altro macroscopico strumento concepito col chiaro intento di penalizzare le produzioni italiane, sottraendo a queste ultime altre importanti quote di mercato. Questo Governo, finalmente, dopo circa un decennio vuole riportare il Paese dalla strada della crisi a quella dello sviluppo e della crescita, valorizzando e riconoscendo la creatività, l'ingegno e la competenza che danno valore ai nostri prodotti. A proposito di questo tema, cui è strettamente collegato, la scorsa settimana abbiamo approvato uno scostamento di bilancio pari a 3,4 miliardi di euro, ieri il Governo ha immediatamente destinato a sostegno del lavoro, di tutti i lavoratori in forza e anche dei disoccupati, perché entrino al più presto nel mondo del lavoro

Presidente, vorrei ricordare a quest'Assemblea un dato che è passato in sordina. Ad aprile 2023 si è stimato un aumento sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori sia dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese. La dinamica positiva riflette il miglioramento dei giudizi sulla situazione economica generale e nasce certamente dalle iniziative che stanno portando avanti il Governo e il Parlamento. È evidente che in quest'Aula

Chi vota contro o chi si astiene su questo provvedimento, vota contro il bene del futuro dell'Italia, delle imprese e degli imprenditori italiani

il disegno di legge in esame modifica il codice della proprietà intellettuale, introduce importanti semplificazioni normative, rafforza la protezione dei marchi,

3, 4 e 5, in cui viene normato il trasferimento della titolarità dell'invenzione industriale dall'inventore (identificato come dipendente) alla istituzione, in questo in questo caso l'università o gli enti di ricerca. Chiaramente noi siamo d'accordo in principio su questo concetto, perché è giusto che i risultati di una ricerca realizzata con fondi pubblici in istituti e università pubblici in qualche modo ritornino alla collettività. Tuttavia, a nostro avviso, questo disegno di legge contiene delle ambiguità; in modo particolare, non valorizza il contributo degli studenti e, cosa ancora peggiore, ne ignora le esigenze formative. valorizzazione, gli studenti sono la componente più creativa, ma allo stesso tempo più vulnerabile delle nostre università e dei nostri centri di ricerca. Spessissimo hanno hanno contribuito o contribuiscono all'invenzione industriale e figurano tra gli autori di brevetti, dando quindi un contributo fondamentale. Gli studenti, però, non sono dipendenti: pagano le tasse, eppure in questo provvedimento sono equiparati ai dipendenti. A nostro avviso, le disposizioni che si applicano ai dipendenti non si dovrebbero applicare agli studenti, ai quali dovrebbe rimanere la titolarità per la loro quota parte. Questo ne aumenterebbe la forza contrattuale e le opportunità una volta lasciata l'università. Invece, all'articolo 5, gli atenei e gli enti di ricerca disciplinano nella propria autonomia e tutte le disposizioni di questo disegno di legge si applicano ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, inclusi gli studenti del corso di laurea. Ciò tradotto significa che ogni università, in propria autonomia, decide come distribuire i benefici dell'invenzione industriale agli studenti, a nostro avviso privandoli del diritto di proprietà, in quanto non dipendenti.

di non pubblicare una scoperta scientifica, ne trae un danno grave. Questa legge crea le condizioni proprio perché ciò accada. La concessione della domanda di brevetto, signor Presidente, dipende fondamentalmente da due criteri: l'inventività e l'innovazione. La seconda dipende direttamente dal concetto di priorità, cioè non devono essere disponibili informazioni precedenti che svelino aspetti cruciali dell'invenzione. L'esigenza della priorità - e di questo non ci siamo resi conto - è in conflitto con quella degli studenti di presentare la tesi tempestivamente e quindi completare il corso degli studi e pubblicare i risultati della ricerca. Il disegno di legge concede all'università nove mesi per esercitare l'opzione per presentare la domanda di brevetto, un periodo lunghissimo per uno studente: un laureando può tranquillamente rimandare la laurea, ma un dottorando deve completare in tre anni, e nove mesi sono il 25 per cento del suo tempo.

nel caso in cui l'università non optasse per la protezione dell'invenzione industriale, nulla è previsto per quanto riguarda i tempi che il ricercatore deve utilizzare per presentare la domanda, mettendo quindi lo studente in una situazione di completa dipendenza e incertezza. Nulla è previsto, inoltre, nel caso in cui, una volta che l'università abbia esercitato l'opzione, per qualche ragione non decida di proseguire oltre la fase nazionale e andare a quella europea. La domanda che ci poniamo è cosa accade di questa proprietà intellettuale, a chi ritorna e chi ne è il titolare. Questo, fra l'altro, non è un caso unico: in Italia ci sono 11.000 domande di brevetto e soltanto 4.900 lo scorso anno sono andate al brevetto europeo; ciò significa che 6.000 domande vengono depositate e non proseguono l'*iter*, quindi bisogna chiarire anche questo aspetto. L'ultimo articolo, poi, non prevede alcun finanziamento per l'attuazione di questo disegno di legge. Ebbene, se si trasferisce la titolarità, si trasferiscono anche gli oneri legati alla domanda di deposito dei brevetti. Sono state fatte tante audizioni, ma non ci è stato detto quanto costa un brevetto. Ve lo dico io: passando dall'Italia all'Europa, sono circa 12.000 euro a brevetto, dopo tre anni sono 50.000. Si tratta di costi importantissimi, che le università, allo stato attuale, evidentemente non sono in grado di affrontare. È prevista l'istituzione di un ufficio di trasferimento tecnologico con risorse proprie: ma, signori, un ufficio di trasferimento tecnologico è una cosa seria, ha bisogno di competenze finanziarie e tecnico-scientifiche, nonché di conoscenze del mondo finanziario e industriale. Penso, insomma, che questo provvedimento contenga molti aspetti velleitari. Signor Presidente, le nostre università e i nostri centri di ricerca operano in Italia, non nel Paese delle meraviglie di Alice, dove sogni e desideri non obbediscono alle leggi della fisica e dell'economia.

Lo votiamo oggi dopo ben diciotto anni, ovvero dall'istituzione del codice sulla proprietà industriale risalente al 10 febbraio 2005. Questa normativa viene finalmente aggiornata alle dinamiche e alle logiche industriali dei nostri tempi. La protezione della proprietà industriale e il conseguente rafforzamento della competitività del sistema Paese sono due delle basi su cui il testo si fonda. L'obiettivo sono la semplificazione delle procedure amministrative e la loro digitalizzazione. In questo In questo settore non siamo all'avanguardia: ringraziamo perciò il Governo - il Ministero dell'industria e del *made in Italy* e il suo ministro Urso - che con questa normativa ci allinea ad altri *partner* europei, che già possono fare affidamento su un contesto molto più agile e snello riguardo alla tutela della proprietà industriale. Questo provvedimento va inquadrato in quella serie di atti che, come anche l'Istat ha certificato pochi giorni fa, ci consentono di accelerare sulla crescita e di compiere addirittura un sorpasso su molti Paesi europei, non da ultimo la Germania, la cui economia ristagna da alcuni mesi. Ricordo che il primo trimestre

Le numerose audizioni svolte ci hanno dato preziose indicazioni, da cui abbiamo tratto profitto, e ben sappiamo che queste modifiche al codice della proprietà industriale erano molto attese da tutta l'industria italiana, soprattutto da quella più performante, che fa della ricerca e dello sviluppo il suo fiore all'occhiello, un buon viatico per la messa a terra più snella e veloce di tantissimi progetti del PNRR. C'è un'alta densità di diritti di proprietà intellettuale, che generano oltre il 52 per cento dei PIL nazionale e contribuiscono al 28 per cento dell'occupazione, con risultati migliori della media europea. La stessa Confindustria ha definito in audizione questo disegno di legge una pietra miliare del PNRR, auspicandone una celere approvazione, cui tra poco procederemo. tratta di un mattone importante nella costruzione di un Paese con meno burocrazia, che va resa sostenibile, e di un tassello fondamentale per la difesa della creatività e dell'ingegno del nostro *made in Italy*. Dobbiamo recepire l'insegnamento di Adriano Olivetti e concretizzare quell'umanesimo industriale che prende una cellula di comunità, che è l'azienda, e ne fa società; per farlo, però, dobbiamo anche difendere la proprietà industriale delle nostre aziende, per renderle più forti e competitive. Negli ultimi vent'anni, l'investimento in ricerca e sviluppo delle nostre imprese è raddoppiato, passando dallo 0,5 per cento del PIL allo 0,94 per cento. Bisogna però assicurare alle aziende che questo sforzo non sia vanificato da chi non investe in ingegno, creatività, ricerca e sviluppo, ma si limita ad immettere sul mercato prodotti e marchi semplicemente copiati dal nostro *made in Italy*.

registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi di prodotti con indicazione geografica o a denominazione di origine protetta (IGP e DOP). In questo senso, è importante sottolineare l'introduzione dell'articolo 34-*bis*, che anticipa la protezione dei disegni o modelli esposti per la prima volta in contesti fieristici, nazionali o internazionali, ufficialmente riconosciuti. Ciò significa esporre prototipi frutto di investimenti in research and development (R&D) senza il timore che gli stessi possano essere copiati, vanificando anni di sacrifici e investimenti delle aziende che li espongono. In questa stessa ottica va letto anche l'articolo 20 che, abrogando il comma 3 dell'articolo 129 del codice di proprietà industriale, garantisce una più efficace azione repressiva e una maggiore speditezza. fino ad oggi, in caso di contraffazione su prodotti esposti in fiera, le Forze dell'ordine potevano solo rilevare un verbale; oggi, grazie a quest'abrogazione, possono procedere al sequestro immediato del materiale contraffatto. Il mercato dell'*italian sounding* agroalimentare vale 120 miliardi (la fonte è «Il Sole 24 Ore»). Per fare un paragone, l'*export* italiano nello stesso settore vale la metà, cioè 60 miliardi. Un ulteriore auspicio è che, attraverso questo disegno di legge, l'Unione europea si determini a dichiarare la non conformità di prodotti che imitano le eccellenze e le specialità italiane, fermando sul nascere queste iniziative, che incidono su mercati strategici per i prodotti italiani. Le imprese italiane non possono, non devono e non vogliono competere con aziende sleali che mettono sul mercato prodotti camuffati con un falso *made in Italy*,

Ogni azienda deve occupare il tempo di un suo collaboratore dai 45 ai 190 giorni per l'espletamento delle incombenze burocratiche e servono da uno a cinque anni per il rilascio delle autorizzazioni, solo perché atti e procedure non sono digitalizzati o perché, come spesso accade, chi deve leggere questi atti non è qualificato a trattare gli allegati tecnici. Per le imprese si tratta di una batosta da 57 miliardi l'anno e tutto ciò limita fortemente la competitività. Come dicevo, questo disegno di legge è il primo mattone verso gli obiettivi fondamentali per l'economia del nostro Paese: meno burocrazia e maggiore difesa del nostro *made in Italy*. Dobbiamo continuare a migliorare e questa è la direzione giusta per facilitare a tutte le imprese l'accesso ai beni *intangible*. *(Applausi)*. L'armocromia di questo disegno di legge è quella giusta: il verde, il bianco e il rosso, i colori del nostro *made in Italy*, che questo provvedimento protegge. *(Applausi)*. Per questi motivi, con grande soddisfazione da senatore e - se me lo consentite - anche da industriale, annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia.

il disegno di legge in esame, n. 536, è stato approvato in un testo unificato dalla Camera dei deputati, trasmesso al Senato e assegnato all'8a Commissione, che ha ritenuto, esaminandolo congiuntamente ad altri due disegni di legge presentati in Senato con analogo contenuto, di adottarlo come testo base. Sostanzialmente, per la settima legislatura viene istituita una Commissione bicamerale per il contrasto delle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, in questo caso con un ampliamento di competenze e di materie trattate uno strumento che ovviamente si è evoluto, quello di questa Commissione bicamerale, anche in relazione ai mutamenti normativi e sociali sul tema, che sono stati davvero rilevanti negli ultimi anni. In particolar modo, proprio nell'ottica di questo adeguamento e ampliamento,

La Commissione dovrà individuare le connessioni fra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali e tra le diverse Regioni. Rispetto a quanto previsto in passato, in questo caso si dovrà tener conto del divario nella dotazione di impianti e del traffico dei rifiuti verso le isole. Un'altra competenza prevista dall'articolo 1 è quella di individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazione estere. Qui vi è una precisazione nuova rispetto ai passati compiti della Commissione: tra gli obiettivi delle indagini è compreso anche l'accertamento dell'esistenza e dell'ubicazione degli impianti a cui i rifiuti sono destinati. Altra competenza prevista dall'articolo 1 è quella di verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti. Anche qui vi è una nuova ed integrata competenza, quella di fare questo esame anche in riferimento all'utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in campo ambientale. Si dovrà poi verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinanti e alle attività di bonifica, nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi. Rispetto a quanto previsto in passato, anche qui si ampliano le competenze, ricomprendendo esplicitamente, tra i siti inquinati, anche gli impianti minerari dismessi, e si precisa che la verifica della sussistenza di attività illecite è svolta anche ai fini di individuare il responsabile della contaminazione. Altro tema è quello di verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato, con riferimento alla gestione degli impianti di depurazione delle acque o smaltimento dei fanghi e al trattamento dei gessi. compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi e visite presso gli impianti, in particolar modo quelli che adottano procedimenti innovativi dal punto di vista ambientale o comunque con tecnologie sperimentali e che presentano Alla Commissione sono poi affidati compiti di verifica della corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale e dell'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché d'indagine sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi, diffuso in molte aree urbane e periferiche, come i cosiddetti roghi tossici, e su altre condotte illecite che riguardino gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ovvero i siti abusivi discarica. Tra i nuovi compiti attribuiti alla Commissione, rientra quello di indagare sull'esistenza di eventuali illeciti connessi

ed al suo smaltimento. Questo è sicuramente un tema nuovo, adeguato anche all'evoluzione della materia. Altri nuovi compiti molto importanti sono quelli di indagare in particolar modo sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, commesse anche attraverso sofisticazione e contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettatura e di marchi di tutela, compreso il loro traffico transfrontaliero. Ciò anche al fine di aggiornare e potenziare la normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente, nonché di contrastare il traffico illecito di prodotti con marchio *made in Italy* contraffatti o alterati. Altro nuovo compito è quello di analizzare le cause dell'abbandono sul suolo e nell'ambiente di prodotti monouso, anche, ma non solo, in plastica verificare l'attuazione data alle disposizioni che recano misure sanzionatorie applicabili a tale condotta e proporre iniziative per la promozione dell'uso di prodotti riutilizzabili compostabili o rinnovabili. Infine, sempre con riferimento alle nuove competenze, vi è quella di indagare sulle attività illecite legate al fenomeno delle zoomafie, nonché di verificare la corretta applicazione del titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale, che appunto riguarda il contrasto a queste attività. Il comma 2 prevede che la Commissione, come già avveniva, riferisca alle Camere con relazioni annuali o ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori. Inoltre, dispone che la Commissione possa redigere relazioni speciali su singole tematiche in materia di ciclo dei rifiuti, anche con riferimento alla situazione emergenziale di talune aree del territorio, con riguardo alla gestione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e radioattivi. Il comma 3, un punto molto importante, prevede che la Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. determina l'importanza e il fatto che i suoi poteri siano molto ampi e possano essere molto efficaci. L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, prevedendo 18 senatori e 18 deputati, nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza, in proporzione al numero dei dei componenti dei Gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun Gruppo esistente alla Camera e di almeno un senatore per ciascun Gruppo esistente al Senato. Esso prevede, inoltre, che i componenti siano nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione e che essa sia rinnovata dopo il primo biennio. Detta, inoltre, le norme per il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza. Gli articoli da 3 a 6 sono quelli relativi all'organizzazione ed al funzionamento della Commissione. L'articolo 3 individua gli articoli del codice penale da applicare per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione. L'articolo 4 disciplina l'acquisizione di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché di copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. L'articolo 5 reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto per i componenti della Commissione e per il personale addetto. L'articolo 6 disciplina invece l'organizzazione interna e determina i limiti di spesa e la possibilità di incrementarla con un provvedimento motivato. L'articolo 7 fissa infine l'entrata in vigore del provvedimento al giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. In conclusione, Signor Presidente, ci dotiamo oggi di uno strumento importante di lotta a tutte le mafie che lucrano su un tema che riguarda la salute e la qualità della vita dei cittadini, sul quale è quindi ancora più odioso ogni tipo di infiltrazione criminale e mafiosa. Lo facciamo quindi mettendo in campo una Commissione con poteri più ampi e con nuove competenze in settori strategici come quello agricolo ed agroalimentare, con l'auspicio che ci sia ovviamente un largo consenso e che questo strumento ci aiuti e aiuti tutto il Parlamento a combattere e contrastare in modo unitario unitario ogni forma di infiltrazione mafiosa nelle istituzioni e nel settore industriale e produttivo della nostra Nazione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'istituzione anche nella presente legislatura di una Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti costituisce un passo importante per la lotta alle ecomafie, da condividere a prescindere dalle logiche di appartenenza. I poteri assegnati alla Commissione attengono ad ambiti particolarmente delicati, molto sentiti dall'opinione pubblica, oltre che dalle istituzioni, e vanno nella direzione di rafforzare il doveroso monitoraggio delle regole ambientali e di verificare le attività illecite che spesso contraddistinguono tali settori, peraltro in un contesto come quello attuale, caratterizzato da importanti investimenti nell'ambito delle misure già introdotte dal Governo in questi mesi e degli obiettivi del PNRR. Tali attività, storicamente legate al ciclo dei rifiuti in senso stretto, oggi abbracciano ulteriori campi di azione. Basti pensare al tema dello smaltimento degli impianti di energia da fonte rinnovabile, sempre più rilevante alla luce delle odierne sfide della sicurezza energetica e della necessità di diversificare le fonti energetiche nel delicato contesto geopolitico ed economico internazionale. Parimenti importante è la questione connessa agli illeciti agroalimentari, ai quali è necessario riservare la doverosa attenzione per prevenire e, se necessario, reprimere situazioni di abuso, che possono ledere il peculiare marchio di qualità che da sempre contraddistingue la produzione agricola italiana in tutto il mondo.

Signor Presidente, cari colleghi, sono davvero lieto che in questa legislatura venga istituita la Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali. Sottolineo l'importanza di assicurare la continuità funzionale di un organismo che fu istituito con la legge 10 aprile 1997, n. 97, e che nel corso della XIX legislatura si appresta a celebrare venticinque anni di attività, con l'auspicata concorde approvazione di quest'Assemblea. La tutela della natura, dell'ambiente e del rispetto della filiera del riciclo dei rifiuti è un principio da cui non si dovrebbe prescindere. Abbiamo assistito troppo spesso, in un passato nemmeno troppo remoto, ad intromissioni di varia natura nel sistema dello smaltimento e riciclo dei rifiuti. Noi non vogliamo sostituirci alla magistratura e al suo ruolo nel contrasto malavitoso nel sistema dei rifiuti. Vogliamo essere invece di supporto nello studio del fenomeno criminoso, anche dal punto di vista dell'attività legislativa. L'Italia non può permettersi, sia per rispetto agli italiani di oggi e alle nuove generazioni di domani, sia agli occhi dell'Europa e dei Paesi del G20, oltreché delle Nazioni Unite, di soffrire ancora per il mancato rispetto dei protocolli in essere sull'inquinamento, oltre che per attività illecite nella filiera dei rifiuti. Da medico non posso che condividere e sostenere con convinzione la scelta effettuata da questo Governo e ribadisco il voto favorevole del Gruppo parlamentare Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia)-MAIE a questo provvedimento. *(Applausi)*.

accogliamo con molto favore l'istituzione di questa Commissione, che non consideriamo però un appuntamento rituale di questo Parlamento, anche se è già stata istituita molte volte nel corso delle passate

che hanno a che fare con il ciclo illegale del cemento, ma anche con lo smaltimento abusivo degli inquinanti, fino naturalmente alla corruzione e ai reati contro la fauna. Evidentemente bastano questi dati a darci il segno della necessità di continuare a intervenire su tale questione, che peraltro - come lei potrà immaginare - è molto cara al mio Gruppo parlamentare e alla mia forza politica, che ha fatto del

come ben si capisce, da questo punto di vista è certamente una occasione straordinaria; peraltro, come sappiamo,

Naturalmente dobbiamo impedire in tutti i modi che il PNRR si trasformi in un'occasione per chi specula sulla salute e sull'ambiente. Dobbiamo scongiurare il rischio di penetrazioni e di infiltrazioni ecomafiose nella realizzazione di opere infrastrutturali o nella stessa gestione dei rifiuti, che, come sappiamo, da molti anni a questa parte, è una fonte di reddito particolarmente significativa per le organizzazioni criminali. Peraltro, saluto anche positivamente il dato secondo il quale tra le competenze di questa Commissione vi è anche quella relativa alle agromafie, quindi al controllo e alla gestione - o almeno al tentativo di controllo e di gestione - sempre da parte delle organizzazioni criminali, come per esempio la camorra nella mia Regione, delle filiere agroalimentari dei mercati ortofrutticoli. Anche questo ovviamente è un tema di primaria grandezza. Sappiamo anche - perché ne abbiamo discusso più volte all'interno di quest'Aula anche su altri provvedimenti - che le cosiddette agromafie non si limitano semplicemente a questo, ma per ma per la raccolta dei prodotti spesso utilizzano attività che si collegano al caporalato, quindi anche allo sfruttamento disumano di persone in una particolare condizione di debolezza,

di azione di questa Commissione, includendo, oltre alle questioni che erano già oggetto di attenzione della Commissione nella scorsa legislatura, anche l'attività d'indagine sull'illecito sfruttamento degli animali. Si tratta anche in questo caso di un tema di cui si discute poco, ma assolutamente significativo, che peraltro ha dimensioni molto grandi sia sul territorio nazionale sia sia su quello europeo. È un vero e proprio giro di affari milionari - quello che riguarda, per l'appunto, lo sfruttamento degli animali - addirittura secondo soltanto alla droga e alle armi. Pensate, per esempio, che i cani utilizzati in attività

mettere l'accento - dal nostro punto di vista, molto positivamente - come pure l'articolo 41, sul principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi; anche da questo punto di vista, ci sembra sembra assolutamente pertinente continuare anche in questa legislatura il lavoro che è già stato fatto negli anni passati. Concludo, ribadendo il nostro voto favorevole.

il codice dell'ambiente e la sua rivisitazione, in cui abbiamo introdotto il disastro ambientale, l'individuazione di un deposito unico per i rifiuti radioattivi e la vigilanza dei siti

Ovviamente, grazie all'importanza che ha la transizione ecologica, grazie al PNRR, grazie ai fondi europei, grazie al rilievo che l'ambiente ha nel futuro delle politiche di ogni Stato, è giusto che questa Commissione ampli il proprio raggio di azione. Deve farlo nei confronti delle terre rare, come ha detto giustamente il relatore quando ha parlato dei rifiuti che verranno prodotti dalla transizione ecologica, da

al *made in Italy* agroalimentare che ci rende famosi in tutto il mondo e che, proprio per questo, viene imitato, non soltanto da Paesi stranieri: il più grande Paese che imita i nostri prodotti agroalimentari è l'Australia, il secondo gli Stati Uniti, il terzo il Canada. Si tratta, che hanno una propria legalità e non si parla di criminalità; ma vi è anche la criminalità che decide di speculare e di risparmiare sui

quello di Roberto Saviano - la criminalità organizzata è servita quasi a dire agli imprenditori: smaltiamo noi rifiuti, lo facciamo in modo semplice. Questo deve essere un monito per noi legislatori che, quando facciamo le norme, con tutte le cautele del caso, dobbiamo farle semplici, altrimenti c'è qualcuno che semplifica la vita a chi deve intraprendere l'attività economica.

si è fatta carico di risolvere i problemi di cittadini, soprattutto in quella parte del Paese dove lo Stato appare molto lontano. Non credo che questa Commissione bicamerale abbia un colore politico - per fortuna

criminale e su un ciclo dei rifiuti che deve essere virtuoso. Al riguardo mi piace invece esaltare quei cicli di rifiuti che noi sappiamo fare. Noi siamo *leader* dell'economia circolare, il nostro Paese lo è per quanto riguarda le materie prime seconde. Proprio per chi fa bene il proprio lavoro e per chi ci rende orgogliosi di avere già anticipatamente raggiunto quegli obiettivi previsti dalle direttive nel 2025 e 2030, dobbiamo far luce su chi invece così trasparente e

Si tratta di una filiera assai delicata e sensibile e in questo momento storico assume grande importanza l'intero ciclo dei rifiuti, anche perché ormai, anziché rifiuti, dovremmo chiamarli risorse. La crisi energetica ha mostrato ancora di più come possa essere conveniente la trasformazione di ogni tipo di rifiuto: innanzitutto quelli da inserire nel circolo virtuoso del riciclo, ma anche quelli che possono essere valorizzati e trasformati in energia. Certamente il lavoro della nuova Commissione non parte da zero, posto che questo tipo di Commissione venne istituita dalla XII legislatura. L'ultima Commissione, quella della scorsa legislatura, ha terminato il proprio lavoro nel settembre scorso, con un raggio di azione molto ampio, investigando molti aspetti legati al ciclo dei rifiuti e non solo in Italia. C'è un lavoro da portare avanti, testimoniato anche dalla relazione finale presentata al termine della scorsa legislatura. Per questo vediamo con favore la ricostituzione nell'attuale legislatura che avrà compiti ulteriori e un ventaglio di ambiti da controllare e investigare adeguato alle nuove esigenze. Gli interessi sulla gestione dei rifiuti sono innanzitutto imprenditoriali e su questo tipo di attività ha messo da tempo le proprie mani la criminalità organizzata. Questa è un'ottima ragione per cui è necessario che vi sia un'apposita Commissione che continui a lavorare su questi temi perché, oltre alle tradizionali attività di gestione illecita dei rifiuti, le mafie si insinuano anche in attività di gestione dei cicli successivi. La sola gestione dei rifiuti è un'attività che ha un valore che ormai supera i 13 miliardi di euro all'anno, mentre l'economia circolare vale fino a 100 miliardi di euro solo in Italia. La Commissione dovrà anche tenere conto del percorso verso un'economia sempre più verde intrapreso dall'Unione europea, un percorso che peraltro vincola molte delle scelte che stiamo adottando con il PNRR. La Missione 2, che prevede la rivoluzione verde e la transizione ecologica, ha a disposizione circa 70 miliardi, un terzo del totale. Lo scopo è quello di migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e rendere virtuoso il paradigma dell'economia circolare. Infatti, in quei fondi si prevede la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, prevedendo il miglioramento della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e la realizzazione di nuovi impianti di trattamento e riciclaggio dei rifiuti. Sono previsti anche i cosiddetti progetti faro di economia circolare, le isole verdi, le *green community*. A sostegno di queste misure è previsto un sistema di monitoraggio su tutto il territorio nazionale che consentirà di affrontare tematiche di scarichi illegali, attraverso l'impiego di satelliti, droni e tecnologie a intelligenza artificiale. Si prevedono anche lo sviluppo della logistica per il settore agroalimentare, anche per ridurre gli sprechi alimentari, e il parco agrisolare, cioè l'installazione di pannelli a energia solare, realizzando contestualmente una riqualificazione delle strutture produttive, con la rimozione dell'eternit o dell'amianto sui tetti. Questi 70 miliardi, questi lavori questi fondi fanno gola evidentemente alle ecomafie ed ecco perché è utile l'istituzione di questa Commissione su tutti i temi affrontati, che riguardano l'agricoltura sostenibile, l'economia circolare, la transizione ed efficienza energetica, anche degli edifici, la mobilità sostenibile, le risorse idriche e l'inquinamento. Sono tutti temi che hanno a che fare con i rifiuti e spesso con nuovi tipi di rifiuti. Ad esempio, con le auto elettriche ci sarà una minore emissione di *greenhouse gas*, ma sorgerà il problema dello smaltimento di un maggior quantitativo e un volume più grande di batterie a fine ciclo. ciclo. La stessa coibentazione degli edifici, ancora, non è di durata infinita; periodicamente va sostituita e crea grandi quantità di rifiuti da smaltire. Per questo, dunque, considerato il complesso delle sfide che ci attendono, si rende fondamentale istituire la Commissione, che avrà compiti ulteriori rispetto a quelli delle scorse legislature.

aver avuto la possibilità di mettere in pratica l'attività della Commissione. Perciò posso portare un'esperienza diretta e posso affermare con grande determinazione che la Commissione bicamerale, la cui istituzione ci apprestiamo ad approvare nuovamente, anche per i compiti ulteriori che le vengono assegnati, potrà dare un aiuto concreto al Parlamento, al Governo e alla Nazione. I temi ambientali sono oltremodo attuali e tutto ciò che è correlato ai grandi investimenti economici, ai *business* è di interesse proprio della criminalità e delle mafie.

in una sinergia proattiva. Da parte mia, posso rappresentare che nella passata legislatura la Commissione bicamerale ha avuto un approccio

perciò insieme porteremo nuovamente, in questa XIX legislatura, qualcosa che ci unisce e ci accomuna come la difesa di un bene che è stato inserito in Costituzione. Ricordo ai colleghi che erano insieme a noi che abbiamo approvato quella modifica all'articolo 9, aggiungendo al terzo comma delle precise indicazioni. Questo rafforza il valore di questa Commissione, perciò parliamo di tutela degli ecosistemi e della salute, che è intrinsecamente collegata alla difesa dei beni ambientali. Un'altra modifica costituzionale è stata apportata all'articolo 41 e mi permetto di sottolineare che è stato ben messo in evidenza che ogni attività economica privata non può prevaricare un bene superiore, cioè l'ambiente e la salute che era già in Costituzione e che viene ribadito ulteriormente. ulteriormente. A livello nazionale, ma anche a livello di Unione europea, questo è stato da anni declinato e messo in evidenza. Ci sono tante direttive e regolamenti comunitari che ce lo ricordano continuamente e anche nelle norme nazionali abbiamo trasfuso quello che è un obiettivo delle 27 Nazioni dell'Unione europea. I temi ambientali sono al centro delle politiche nazionali, dell'Unione europea e del mio Gruppo politico, perché il MoVimento 5 Stelle da sempre ha avuto tra le proprie stelle quelle della difesa dell'ambiente. *(Applausi)*. Il faro che ci ha governato da sempre e continuerà a farlo è la difesa degli ecosistemi, dell'ambiente, dell'acqua e della salute dei cittadini, quindi non possiamo che essere favorevoli alla lotta incondizionata a tutte le mafie, nella difesa dell'ambiente e pertanto voteremo a favore di questo importante disegno di legge.

valori che sono assolutamente comuni. Cerco proprio di riprendere alcune delle parole che sono state dette per confortare sicuramente quelle intenzioni che ognuno dei membri della Commissione sarà sicuramente propenso a portare all'interno del consesso che rappresenterà un gruppo di lavoro a favore della nostra comunità e dell'ambiente. Lo si è ricordato poco fa: la modifica costituzionale che ha elevato al rango di obiettivi primari la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è uno dei momenti che credo abbia permesso l'ampliamento delle competenze di questa Commissione. lo diceva poco fa un collega - l'articolo 41 a proposito dell'obbligo che vige per le attività economiche pubbliche e private, e che adesso è diventato norma di rango costituzionale, di rispettare nell'ambito delle attività produttive e della produzione di beni e servizi quell'ambiente che, purtroppo, fino ad oggi non siamo riusciti a preservare preservare da indegne condotte che diventano debiti per le generazioni future. Quando si fanno indagini su avvenimenti e fatti, bisogna anche capire qual è la logica che spinge questo tipo di *business* a continuare a perpetrare i propri effetti nefasti sulla nostra comunità. Voglio solo ricordare cosa c'è dietro a questo *business*. Evidentemente c'è anche la cultura dei no; quella cultura che, purtroppo, spesso e volentieri costringe amministrazioni comunali come Roma capitale a dover spendere 180.000 euro a settimana per trasportare dei rifiuti in Olanda. Ebbene, pensate quanto

questa Commissione di inchiesta dovrà cercare di capire come mai fino ad oggi il termine "risorsa" l'abbia utilizzato la criminalità organizzata e non la pubblica amministrazione *(Applausi)*, magari costruendo impiantistiche utili a fare redditività a favore della comunità.

si tratta delle garanzie che anche nel *post mortem* sono in grado di preservare la comunità dai debiti, visto che purtroppo molto spesso ci ritroviamo a dover stanziare dei fondi. Lo dico direttamente

cose che a volte ci sono un po' estranee - e che naturalmente hanno alla base il principio della correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente, semplicemente l'applicazione del principio "chi inquina paga".

approvare le importanti relazioni che costituiranno fattor comune di questa Assemblea parlamentare, per renderla edotta dei tanti segreti e trucchi

può costare da 200 a 250 euro, la spesa illegale si attesta invece sui 100-150 euro. Per risolvere il problema ci vogliono tecnologie e impiantistiche e occorre dare spazio a quelle virtuose esperienze che è giusto che entrino anche all'interno delle strutture della pubblica amministrazione, con collaborazioni e arricchiscano il patrimonio professionale dei soggetti deputati a prendere decisioni pubbliche nell'interesse della collettività.

Il fatto che lo si faccia unanimemente è un segnale positivo, così come è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento. Ed è un auspicio per rafforzare un impegno comune contro la criminalità; un impegno che consenta di riaffermare, partendo dalle istituzioni, l'esigenza di una diffusa e coerente pratica della legalità. Ci auguriamo - lo dico subito, Presidente - che questa deliberazione unanime trovi le gambe per camminare camminare e che i Presidenti di Camera e Senato, sollecitando le designazioni dei membri da parte dei Gruppi, possano al più presto istituire la Commissione. Sottolineiamo questo perché dal 2 marzo scorso le Camere hanno approvato la legge istitutiva della Commissione parlamentare antimafia e da allora ne attendiamo la costituzione. *(Applausi)*. È un ritardo grave, perché la mafia è tutt'altro che sconfitta nel nostro Paese. Gli appetiti criminali si fanno sempre più forti, a fronte delle ingenti risorse che giungono, che sono giunte e stanno giungendo nel Paese. Avere quindi la Commissione antimafia operativa significa poter aiutare a leggere con attenzione tutto ciò che sta avvenendo nei territori, nel Paese e capire come intervenire e coadiuvare gli sforzi della magistratura e delle Forze dell'ordine per contrastare la morsa degli interessi mafiosi e delle troppe connivenze che ancora li sostengono. A questo proposito mi sia consentito dire, pur in un clima che giudichiamo positivamente, che consideriamo un errore grave, in questo quadro, avere indebolito per esempio il codice degli appalti e aver alzato il tetto dell'uso del contante. *(Applausi)*. Ci auguriamo che questo ritardo venga recuperato con immediatezza, unitamente all'avvio di questa Commissione. Ad allarmare e a rendere urgente l'inizio dei lavori della Commissione che istituiremo a breve stasera stanno anche i recenti dati allarmanti che Legambiente ha diffuso Oggi - come è stato ricordato già da altri intervenuti - abbiamo dei motivi in più, perché questo Parlamento ha messo in Costituzione, nel suo articolo 9, il principio della tutela dell'ambiente. Così come altrettanto significativo è stato aver modificato l'articolo 41, 41, mettendo bene in rilievo che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti che riguardano la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Sono segnali tra l'altro inequivocabili di prospettiva del nostro Paese e della necessità di avviare con compiutezza la fase della transizione ecologica, fino ad arrivare all'obiettivo dell'uscita dall'era dei combustibili fossili e alle alle emissioni zero entro il 2050. Su questo abbiamo accumulato gravissimi ritardi - diciamolo - anche rispetto a direttive e impegni europei; ritardi che - secondo noi - vanno rapidamente colmati, con coraggio e senza tirare il freno a mano davanti a decisioni europee che vanno nella direzione di

Fin dall'inizio, dalla sua prima istituzione durante la XII legislatura, ha rappresentato un punto di osservazione e di iniziativa molto qualificato e di controllo su un tema obiettivamente complesso,

un insieme di misure legislative nei confronti degli ecoreati. Quello fu uno dei punti più qualificanti di quella legislatura: l'approvazione di quella legislazione in materia di tutela ambientale contro i reati ambientali. Noi dobbiamo andare in questa direzione non solo contrastando penalmente i reati - cosa che dobbiamo fare e che la Commissione aiuterà a fare - ma anche e soprattutto con uno sviluppo dell'economia circolare, che è un ambito strategico, dove stanno insieme protezione dell'ambiente, qualità della vita e sviluppo economico. Noi abbiamo una percentuale di riciclaggio davvero pesante. In alcune aree del Paese c'è un riciclaggio dei rifiuti molto avanzato, ma in alcune altre

la posizione di *leadership* dell'Italia nell'economia circolare, area nella quale già possiamo vantare una eccellenza. All'interno di questa prospettiva vi sono, però, dei dati allarmanti. Mi riferisco al rapporto di Legambiente. Nel 2021 i reati contro l'ambiente non scendono sotto il muro dei 30.000 illeciti: 30.590 illeciti, 84 reati al giorno, 3,5 ogni ora; quasi 60.000 gli illeciti amministrativi contestati; 115 sono state le inchieste su corruzione da parte della magistratura; 14 i Comuni sciolti per mafia nel 2021 e 7 nel 2022. Le inchieste contro i traffici illeciti di rifiuti monitorate da Legambiente nel 2021 sono state 38 contro le 27 dell'anno precedente e sono andati in aumento i reati. Perfino il traffico illecito degli oli vegetali esausti ha conosciuto un aumento. Insomma, sono i dati a raccontarci di un Paese ancora segnato pesantemente dalla criminalità ambientale, che assume anche forme diverse da quelle del passato e che necessitano, quindi, di analisi aggiornate e di strumenti assolutamente adeguati, per poter meglio prevenirle e contrastarle.

Le inchieste e le relazioni hanno riguardato e hanno acceso luci importanti su fenomeni quali il traffico transfrontaliero dei rifiuti; lo stato di attuazione delle bonifiche nei siti di interesse nazionale; la gestione dei rifiuti radioattivi; la realizzazione del deposito unico nazionale; il tema degli incendi negli impianti di rifiuti, senza contare l'approfondimento e le due relazioni approvate sulle garanzie finanziarie nel settore delle discariche, modo come i fenomeni di illegalità ambientale spesso sono connessi ad aspetti finanziari e organizzativi del ciclo di gestione dei rifiuti. Insomma, signor Presidente, l'Italia ha già pagato per non avere rispettato la tutela dell'ambiente, per avere spesso cementificato e per avere enormi difficoltà anche nell'abbattimento degli abusi edilizi. Ha pagato prezzi altissimi. Il nostro territorio ha scarsa qualità di opere, che poi alla fine non reggono davanti alle calamità naturali. L'assetto e il rammendo del territorio non ci sono stati, nonostante gli sforzi anche dei Governi passati. Questo prezzo che l'Italia ha pagato ora pesa su di noi ed è per questo che dobbiamo prevedere per le future generazioni, per oggi e per domani, un cambio di marcia. Servono il sostegno dello Stato alle pubbliche amministrazioni e procedure tecnologicamente avanzate; serve rafforzare il sistema dei controlli, approvando i decreti attuativi della legge sul sistema nazionale di protezione ambientale.

il mio capogruppo, Lucio Malan - non è presente - e il mio partito, per avermi scelto per la dichiarazione di voto su un tema a me molto caro, per il quale mi batto da anni. So che dirsi emozionati quando si parla di rifiuti e del mondo degli illeciti ad esso connesso può sembrare strano; ma, in realtà, è proprio la passione che movimenta e anima il mio lavoro da amministratore di professione, che mi porta a mettere

Non parlerò di numeri, perché lo ha già fatto chi mi ha preceduto, ma in questi pochi minuti cercherò di raccontare e sintetizzare quelle azioni che la Commissione dovrà espletare al fine di combattere gli illeciti agroalimentari, gli illeciti ambientali, quelli legati al ciclo dei rifiuti e quelli legati al ciclo dell'acqua. Rivolgo un ringraziamento al relatore, senatore De Priamo, alla Camera

la Commissione parlamentare che - come abbiamo visto - presenta però una dicitura ampliata rispetto a quella del passato. Includere temi quali gli illeciti agroalimentari e gli illeciti ambientali, per iniziativa della maggioranza, fa capire che noi ci siamo e che, fino a oggi, chi ci ha sempre accusato strumentalmente di non essere sensibili alle materie ambientali si sbagliava di grosso. La dimostrazione è ciò che abbiamo fatto integrando il disegno di legge Quindi, signor Presidente, questa Commissione sarà chiamata a fare un salto in avanti rispetto a quello che è stato fatto dal precedente Governo.

poi fare attività di indagine con l'autorità giudiziaria; dare inizio a un'attività vera e propria di ricognizione, con una progettazione per il risanamento dei luoghi monitoraggio successivo del ripristino dei luoghi e della legalità. Infine, abbiamo anche inserito il monitoraggio per verificare come vengono spesi i soldi del PNRR. Questo è ciò che abbiamo detto tutti, per me la Commissione deve andare molto oltre. La Commissione non deve esaurire qui il suo lavoro, ma deve andare a monte dell'illecito e ciò significa capire dove la malavita è riuscita ad insinuarsi in processi così delicati. Per fare ciò occorre lavorare su tre concetti fondamentali: norme e burocrazia, ideologia del no a prescindere ed educazione ambientale, che purtroppo non ho mai sentito nominare oggi, in questi giorni e neanche alla Camera «norme e burocrazia»? Onorevoli colleghi, vi siete mai soffermati a contare e a leggere le norme nazionali che regolamentano la gestione dei rifiuti e delle acque? Migliaia e migliaia di pagine, con frasi a volte incomprensibili, a volte in contrasto tra loro, che si prestano facilmente a interpretazioni soggettive. Questa è solo la punta dell'*iceberg*, perché da qui ha inizio la grande frammentazione delle leggi regionali. Per darvi un'idea: la gestione dei rifiuti a livello italiano? La gestione dei rifiuti viene data in mano alle Regioni; le Regioni, a loro volta, delegano gli ATO, i famosi Ambiti territoriali sono 65 gli ATO in Italia e ognuno è dotato di un proprio regolamento e i regolamenti a volte non parlano tra loro. All'interno della stessa Regione - prendo l'esempio della Toscana - abbiamo tre ATO, che hanno tre regolamenti diversi. *(Applausi)*. Se voglio portare un rifiuto dal mio ambito ad un altro, diventa difficile: devo iniziare a chiedere permessi su permessi e diventa veramente una crociata. In questo ginepraio di leggi, norme e regolamenti, immaginate con quanta facilità la criminalità e le organizzazioni a delinquere riescono a fare breccia. È chiaro che non si può andare avanti così. La lotta agli illeciti passa anche e soprattutto attraverso la presa di coscienza di questo stato dei fatti. Questa Commissione dovrà fornire al Governo materiali utili per definire un impianto normativo che parli una sola lingua per tutto il territorio italiano *(Applausi)* e, soprattutto, sia comprensibile anche ai Paesi frontalieri. Noi portiamo i nostri rifiuti nei Paesi vicini, dove la normativa è completamente diversa, e possono fare un tragitto completamente diverso dal nostro, addirittura con una facilità che a noi sembra veramente utopia: sembra il Paese delle meraviglie. È ancora peggio quando andiamo a portarli in mare, utilizzando le navi. Queste normative tra loro non parlano. Ecco che questa Commissione dovrà fornire al Governo tutti i materiali per far sì che la legge sia unica e capibile da tutti. Altro concetto su cui la Commissione dovrà lavorare è l'ideologia del «no» a prescindere. Ho sentito parlare tanto qui, nelle ultime settimane, ma anche in questi anni, di transizione ecologica, economia circolare e politiche *green* per uno sviluppo sostenibile. Signor Presidente, sono tutte belle locuzioni, bellissime, che piacciono ai colleghi dell'opposizione, soprattutto se c'è qualche inglesismo di mezzo,

Come ho fatto rispettare anche il vostro intervento, chiedo a tutti di rispettare l'intervento della collega. PETRUCCI *(FdI)*. La locuzione «economia circolare» definisce un sistema pensato per potersi rigenerare da solo, garantendo la sua ecosostenibilità (definizione che troviamo su tutti i libri e su Internet), non andando a intaccare le risorse presenti in natura, che serviranno alle future generazioni. Applicando questa definizione al ciclo dei rifiuti in Italia, vediamo che non si completa. I rifiuti prodotti dai cittadini, una volta differenziati, vengono raccolti, inviati agli appositi impianti di riciclo per produrre materie prime seconde, su cui saranno realizzati nuovi oggetti, ma il cerchio per chiudersi ha bisogno che tutte le tipologie di rifiuti raccolte vengano trattate e trasformate in nuovi prodotti: non solo plastica, carta, vetro e alluminio, ma anche il rifiuto indifferenziato, il cosiddetto secco, con cui oggi noi facciamo il combustibile solido secondario (CSS), che serve a produrre energia. Sapete come produce energia? Con gli appositi impianti. L'alternativa è la discarica. Questo cerchio non si chiude qui, Presidente, perché questi impianti in molte Regioni non vengono realizzati. Ecco che si interrompe la famosa economia circolare e si apre un altro spiraglio per le ecomafie. Succede che in alcune Regioni il no ideologico alla realizzazione degli impianti che chiuderebbero il famoso cerchio causa invece un triplice danno: economico, ambientale e illegale. *(Applausi)*. Il rifiuto invece di produrre energia a costo zero, a chilometro zero, con costi contenuti e conseguente abbattimento delle tariffe per i cittadini, prende la strada per mare e per terra verso altre Regioni o - ancora peggio - verso altri europei, come la Bulgaria. Smaltire una tonnellata di CSS costa 200 euro. Lo fa il Comune di Grosseto, che, purtroppo, deve portarlo in Bulgaria perché non ci sono impianti che

Tutto questo determina la nascita di un sistema di gestione aleatorio approvato dall'affollamento delle norme di cui dicevo prima: il *mix* perfetto per la criminalità organizzata. rifiuti. Il terzo e ultimo aspetto che la Commissione dovrà trattare, anche se non rientra nei suoi compiti, è l'educazione ambientale. Una volta acquisiti i dati materiali e i risultati d'indagine, i membri dovranno trasferire questa conoscenza ai cittadini attraverso corsi di informazione e formazione. L'educazione ambientale può essere fatta ovunque e a chiunque senza limiti di età. In un momento come questo in cui le politiche ambientali rappresentano il futuro del Paese *(Commenti)*, dobbiamo giocare un ruolo importante nel diffondere, oltre che le buone pratiche da adottare per preservare il nostro pianeta anche la conoscenza delle realtà delinquenziali rappresentate dalle ecomafie che, proprio nell'ignoranza, trovano terreno fertile. Signor Presidente, colleghi senatori, per questo e per tutte le ragioni e i numeri che abbiamo ascoltato, annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia all'istituzione,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

Alle ore 9,20 del 30 aprile 1982, l'onorevole Pio La Torre, segretario regionale del Partito Comunista, accompagnato dal suo amico autista Rosario Di Salvo, si stava recando nella sede del partito di Corso Calatafimi Quando la macchina si trovava in Piazza Generale Turba, una moto di grossa cilindrata obbligò Di Salvo che guidava a fermarsi immediatamente. Seguirono raffiche di proiettili. Da un'auto scesero altri killer a completare il duplice omicidio. L'onorevole Pio La Torre morì all'istante, mentre Rosario Di Salvo ebbe il tempo di estrarre la pistola e sparare alcuni colpi prima di morire. Fino alla fine cercò di proteggere il suo segretario regionale. Nella storia del nostro Paese era la prima volta che un deputato e segretario regionale del Partito Comunista veniva ucciso in un agguato politico mafioso. L'onorevole Pio La Torre è stato un parlamentare della nostra Repubblica dal 1972 al 30 aprile 1982. anni dal tragico agguato nei suoi confronti e nei confronti di Rosario Di Salvo, ci rendiamo conto che, oltre a ricordarlo e farne memoria, noi siamo chiamati anche e soprattutto a mandarlo a memoria. Così si diceva a scuola per le poesie e così sentiamo di poter dire per una vita esemplare, una testimonianza totalmente spesa per il bene della sua gente di Sicilia e dell'intero Paese. Se qualcuno cerca i patrioti nella nostra Nazione, abbiamo ragione di affermare che l'onorevole Pio La Torre ne costituisce un fulgido esempio. La sua acuta e fine intelligenza, maturata alla luce degli studi e ancora di più nel radicamento delle classi popolari della sua terra, gli hanno consentito di poter capire in profondità e leggere come pochi il fenomeno mafioso e individuare quindi gli strumenti più efficaci per contrastarlo. L'onorevole Pio La Torre ha inteso il suo impegno politico e la politica nella sua interezza come un argine al malaffare, senza compromesso alcuno, senza riguardi, senza indulgenze, anche quando le mafie, laddove si camuffavano, riescono a lusingare, a compiacere, a toccare il tallone d'Achille delle persone e delle istituzioni. Pio La Torre ha individuato piuttosto alcuni punti deboli dell'agire mafioso, che fino a quel momento erano perseguiti e ostentati dai boss come segni di forza: l'accumulo della ricchezza Per questo dico che oggi, con un'attualità bruciante e pressoché urgente, abbiamo bisogno di mandare a memoria la lezione di vita di Pio La Torre. Oggi più che ieri le istituzioni hanno bisogno di affinare conoscenze, informazioni e strumenti per impedire la crescita e la diffusione dell'economia e dei poteri delle mafie che hanno cambiato pelle; sono liquide, hanno occupato spazi nella mente di tante persone, mai affiliate ma culturalmente vicine a quel modo di pensare e di agire. A lui dobbiamo la presentazione nel 1980 di un disegno di legge che introduceva il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e il sequestro e la confisca dei beni dei mafiosi. Il testo, però, diventa legge solo nel settembre del 1982, solo dopo la morte di Pio La Torre e del generale Dalla Chiesa. La sua intelligenza (da *intus legere,* leggere in profondità) gli ha consentito anche di vedere i rischi globali che si mimetizzavano dietro il falso mito della sicurezza e si è opposto con tutta l'energia di cui era capace all'istallazione dei missili a Comiso. La storia e il ricordo di Pio La Torre è una storia di oggi: la storia emblematica di un'Italia che voleva e riusciva a pensare in grande, guardando al futuro; la storia di un Paese che non voleva voltarsi dall'altra parte. Aveva capito già negli anni Settanta che la mafia siciliana si era allargata al Nord, che operava nella finanza e nell'impresa. Appena eletto in Parlamento nel maggio del 1972, entrò a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie. L'introduzione dell'articolo 416-*bis* del codice penale e la legge sulla confisca dei beni mafiosi rappresentano per il nostro Paese uno dei grandi lasciti di Pio La Torre: proposte che segnano una svolta radicale nella lotta contro la criminalità organizzata. Aveva messo insieme le due grandi battaglie di civiltà: l'impegno per la pace e l'impegno contro la mafia. la modernità di un uomo politico che aveva uno sguardo lungo e largo nell'affrontare le questioni della libertà, dell'intimidazione mafiosa che uccideva le persone e lo sviluppo sociale ed economico. L'omicidio dell'onorevole Pio La Torre si inquadra in questo contesto. Tanti erano i segnali che si sono voluti dare al Paese con il suo omicidio, uno tra tutti quello preventivo, proprio per la sua attività contro la mafia: era riuscito a far unificare due disegni di leggi in un unico testo per accelerarne l'approvazione. La mafia e i poteri politici che si nutrivano dei rapporti con la mafia non lo potevano tollerare. L'altro segnale era quello intimidatorio: la politica non doveva occuparsi degli arricchimenti illeciti dei mafiosi e di coloro che con la mafia convivevano e colludevano. Il lascito politico, sociale e civile dell'onorevole Pio La Torre non possiamo e non dobbiamo disperderlo. È un lascito che deve trasformarsi in responsabilità davanti al Paese e che ci riguarda tutti, opposizione e maggioranza. Ha pagato il prezzo più alto: sia una testimonianza per tutte e tutti. Senatrice, le ho lasciato qualche minuto in più, perché non si può zittire la lotta alla mafia e, quindi, la ringrazio. La Presidenza si associa alle sue parole.